Signor Presidente, diceva Oscar Luigi Scalfaro che il Parlamento non è più tale perché non si parla, si legge, ciascuno il proprio testo. Direi che la cosa è andata avanti. Oggi non si ascolta più, si vota e spesso la genesi dei voti è oscura, non viene dichiarata in questa Assemblea, ed è frutto di trattative che si svolgono altrove, in sedi extraparlamentari, e che sono coperte da riserbo, un riserbo immotivato e immotivabile. Per esempio, mi sarei aspettato che ieri pomeriggio, in Aula, qualcuno spiegasse quanto successo durante tutta la giornata: per sei volte una forza politica che fa parte della maggioranza di Governo non ha dato il suo contributo al momento della verifica del numero legale, bloccando i lavori dell'Assemblea. Poi si è presentata. Che cosa ha ottenuto in cambio, durante questa trattativa, facendo pesare la sua assenza? Secondo «il Fatto Quotidiano» avrebbe ottenuto l'impegno del senatore Lumia senatore Lumia a ritirare un emendamento nel quale si prevedeva che i termini della prescrizione per determinati reati ambientali, per esempio quelli da amianto, non scattino più

Altri sostengono che l'oggetto della trattativa oscura di ieri sia stato l'imposizione della fiducia. Non vedo ancora il ministro Boschi, ma può darsi che venga a porre la questione di fiducia. Altri ancora collegano quanto avvenuto con ciò che stava accadendo nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, dove è successo qualcosa di fortemente innovativo: la maggioranza di Governo ha presentato una mozione parlamentare che, a differenza delle altre mozioni parlamentari, che da sempre impegnano il Governo, questa volta impegna il Parlamento a cambiare una legge che detta maggioranza di Governo ha approvato in via definitiva appena pochi mesi fa

di una forza della maggioranza ieri in Senato, sia lo stravolgimento del senso della mozione parlamentare - che umiliano il Parlamento e quando l'umiliazione viene dallo stesso Governo e dalla stessa maggioranza bisognerebbe porsi delle domande. Veniamo al provvedimento che esaminiamo oggi. Dico subito che vi sono molti aspetti di questo provvedimento positivi e migliorativi del codice penale e del codice di procedura penale e do atto al ministro Orlando di essersi impegnato, di esser stato presente in Commissione, di aver tolto dal tavolo alcuni strafalcioni e intralci, ma se voi leggete sul frontespizio il tema del provvedimento già capite che la vera questione del dibattito, quella che sta a cuore a una parte consistente dell'opinione pubblica, viene nascosta, in stile trasformista, perché la maggioranza è disomogenea e quindi ogni volta che si discute di cose serie si divide e per non farla dividere si nasconde la natura del contendere. Vi leggo un brano, se avete la pazienza di ascoltarlo: «In Italia, in prigione forse anche i benestanti, i professionisti, le persone più o meno importanti e quelle che appartengono a una certa a una certa classe sociale ci fanno qualche volta una capatina, ma quanto a restarci ci restano solo i poveracci (...) Novantanove volte su cento, infatti, con il tempo, con gli appelli, i contrappelli e la Cassazione, e la Cassazione, anche le condanne iniziali vengono poi cancellate». Chi ha scritto questa frase? Il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle che ieri abbiamo sentito tuonare in quest'Aula? L'ha scritta un'attivista di «Libera»? No, cari colleghi, questa frase è stata scritta sul «Corriere della Sera» di lunedì

lor signori, noi signori possiamo dire, in carcere non ci andiamo mai, se riusciamo ad evitare la punizione, se qualunque avvocato si trovi davanti un cliente danaroso, prima ancora di vedere il merito

quella che dice che non possiamo continuare così, bisogna dare una giustizia giusta, ad un certo punto, bisogna frenare questa tendenza del ricco e potente a difendersi non nel processo, ma dal processo; quella che dice che non si può mantenere un'accusa a vita nei confronti di un cittadino, e la ragionevole durata del processo è un principio di garanzia assolutamente non eliminabile. Sarebbe stato bellissimo se ci fosse stata una discussione di questo genere. Avrei partecipato. Personalmente, con grande rispetto per i colleghi della destra che hanno sostenuto le tesi più garantiste, tra le due esigenze sostengo che in una situazione eccezionale, in attesa che si renda più veloce la giustizia, si può stabilire che dopo una condanna di primo grado (in realtà, ci sono già due sentenze del giudice terzo, perché c'è anche il gip), i termini di prescrizione si fermino, costringendo l'avvocato dopo la condanna e non prima a difendere l'imputato nel processo e non dal processo, con il cavillo, con la lettera che non arriva, con la *mail* che si perde da qualche parte. Ma questa è la mia posizione, ci sono colleghi che vengono dai ranghi della magistratura o dell'avvocatura che ne sanno molto più di me. Avrei ascoltato con interesse e rispetto il loro punto di vista. Ma non è questa la discussione che si è svolta né in Assemblea e purtroppo neppure in Commissione. La discussione che si è svolta è un'altra. Per esempio, le due anime hanno trovato un'intesa con un espediente un espediente molto popolare, demagogico, qualcuno direbbe populista: aumentando le pene. Nel provvedimento c'è un aumento delle pene per i reati che sono tipici dei colletti bianchi e c'è un aumento, per *par condicio*, anche delle pene per il furto e del furto con strappo. Tra l'altro, l'aumento delle pene significa spesso l'aumento del minimo della pena, che è un'operazione - ne siate coscienti, senatori - che vuole legare le mani al giudice. Questo nega un po' sia il garantismo, sia lo Stato di diritto perché ci sono casi in cui il giudice, se non è vincolato da un minimo di pena molto alto, può riconoscere che quel determinato reato e quella fattispecie non aveva la stessa capacità aveva la stessa capacità di offesa di altri reati che hanno lo stesso titolo ma sono commessi in una situazione diversa. Questo modo di nascondere le contraddizioni che ci sono in una maggioranza - ripeto - trasformista e di fare la faccia feroce all'esterno, in modo che ognuno possa aumentato le pene per i reati contro la pubblica amministrazione e di averle aumentate anche per lo zingaro che fa il furto con strappo, per la zingara che attenta alla vostra proprietà nella metropolitana di Roma, questo modo di fare è un modo che delegittima fortemente il Parlamento. Da questo punto di vista, trovo che il provvedimento che noi discutiamo, pur con degli elementi assolutamente apprezzabili, sia profondamente ambiguo, figlio di una legislatura in cui invece di discutere davvero, di dividersi e poi di trovare sintesi in Parlamento, si cercano altre soluzioni, ripeto, sostanzialmente trasformistiche.

dalla società italiana. Ma la colpa di questo è proprio di coloro i quali, in nome della governabilità, procedono sempre a nuove imposizioni o a rinvii quando le imposizioni non sono possibili. Consiglio agli onorevoli colleghi di leggere l'articolo di Michele di oggi, che spiega come si sia passati dalla rottamazione muscolare, dalla grinta nei confronti delle perdite di tempo e dalla velocità

Signor Presidente, stiamo affrontando una riforma di grande portata. Sono interessati circa quaranta articoli del codice penale e del codice di procedura penale, quindi si tratta della legislazione vigente su temi estremamente delicati. Nel tempo che mi è stato assegnato farò una ricognizione abbastanza puntuale, ancorché per titoli e non analiticamente per ogni articolo, con qualche commento su quello che è stato soprattutto il lavoro della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e, in questo ambito, del Gruppo parlamentare che Gli argomenti del disegno di legge sono vari e riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento dei reati contro il patrimonio, la delega per la riforma delle intercettazioni e varie misure sulla semplificazione del processo penale. Inoltre, è stato affrontato il tema della riforma

riguarda gli articoli dal 7 al 12 del disegno di legge, che concerne la prescrizione. Dopo l'esame della Camera dei deputati sono state attuate due modifiche principali all'attuale disciplina della prescrizione: uno scenario riguarda tutti i reati, il secondo scenario attiene a tre specifici reati. Per tutti i reati, la sospensione della prescrizione di giudizio è di due anni dopo la condanna di primo grado e di un anno dopo l'appello. Una eventuale ulteriore sospensione della prescrizione

Per tre specifici reati si introduce un regime speciale: per la corruzione per l'esercizio della funzione, (articolo 318); per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319); la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*). Il tempo necessario a prescrivere il reato, per questi specifici reati, non sarà più pari soltanto al massimo della pena edittale, ma sarà pari al massimo della pena edittale aumentato della metà. Entrando in un argomento più puntuale, rilevo che, a seguito del lavoro della Commissione e dell'approvazione degli emendamenti del Gruppo di Area Popolare, si riscontrano alcune modifiche, che vado ad elencare. Per tutti i reati, la sospensione del termine di prescrizione risulta di un anno e sei mesi

L'estinzione della prescrizione non sarà più possibile in caso di perizie particolarmente complesse (prima dell'intervento della Commissione giustizia del Senato quest'argomento aveva un lasso temporale di tre mesi) l'istanza di ricusazione del giudice porterà all'estinzione della prescrizione. Il ritiro e la bocciatura di alcuni emendamenti sulla decorrenza della prescrizione dall'acquisizione di notizia di reato e sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sono stati causa di un ricondizionamento del quadro. Per i predetti reati di corruzione viene confermato l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (il massimo della pena aumentato della metà) ma viene esclusa la possibilità che si possano aggiungere a tale calcolo i casi di interruzione della prescrizione. In questo modo, si riduce il tempo massimo per prescrivere: ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari 18 anni invece dei 21 anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera.

per prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per esercizio della funzione (articolo

L'allungamento della prescrizione per tali reati risulta ancora più accentuato considerando che le pene per gli stessi reati sono già state recentemente inasprite dalla legge n. 69 del 2015 (cosiddetta legge Grasso).

157 rispetto all'attuale formulazione del codice penale. Passiamo a fare qualche osservazione sull'articolo 158, che riguarda la decorrenza della prescrizione.

L'esame in Commissione al Senato conferma la modifica della Camera. Andiamo ora alle considerazioni concernenti l'articolo 159, che riguarda la sospensione della prescrizione. dei deputati specifica che il termine da cui la prescrizione è sospesa è quello della data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. specifica anche che il termine è sospeso fino alla definizione del giudizio cui è stata deferita la questione. Vengono inserite poi tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: la rogatoria all'estero, le perizie di particolare complessità

il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno; infine, in caso di assoluzione dell'imputato nel grado successivo di giudizio, i predetti periodi di sospensione vengono ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (per esempio, autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice e assenza dell'imputato) il termine è conseguentemente prolungato. La Commissione del Senato, intervenendo su questo *corpus* legislativo, specifica che, in caso di deferimento della questione ad altro giudizio, il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione. stabilisce che la sospensione della prescrizione non è più prevista in caso di perizie di particolare complessità e di istanza di ricusazione del giudice e modifica gli ulteriori casi della sospensione della prescrizione come segue. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Infine, i periodi di sospensione vengono ricomputati nel determinare il termine di prescrizione, anche nel caso in cui la sentenza sia dichiarata nulla, ai sensi dell'articolo 604,

a qualche commento riguardante l'interruzione della prescrizione, regolata all'articolo 160 del codice penale. La Commissione del Senato conferma il testo approvato con cui si precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero determina l'interruzione del corso della prescrizione, superando una questione di carattere interpretativo sorta in casi particolarmente in casi particolarmente frequenti nella giurisprudenza. Svolgo ora qualche riflessione sugli effetti della sospensione e dell'interruzione (parliamo dell'articolo 161 del codice penale). dei deputati prevede che l'interruzione abbia effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. La formulazione vigente del codice penale dispone che tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso un reato. giustizia del Senato conferma quanto disposto dal testo della Camera riguardo agli effetti differenziati di interruzione e sospensione: conferma l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (massimo della pena aumentato della metà), ma, modificando il riferimento normativo rispetto al testo della Camera, esattamente dall'articolo 157 all'articolo 161 del codice penale, consente di ricomprendere nell'aumento dei tempi di prescrizione anche gli atti interruttori. In questo modo si riduce il tempo massimo per prescrivere. Ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 saranno necessari diciotto anni invece di ventuno anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita, dare o promettere utilità (articolo

e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*). Questi interventi, come gli altri che ho precedentemente citato, votati a larga maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, sono emendamenti proposti dal Gruppo Area Popolare. disciplina delle notificazioni, che può sembrare un argomento quasi di ragioneria del diritto, una *technicality*, ma ha notevoli conseguenze sul diritto alla difesa e sull'intero *iter* processuale, anche in termini di sostanza. Il ritiro dell'emendamento dei relatori, il 16.0.1000, che riscriveva l'intera materia delle notificazioni con una finalità acceleratoria che non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, metteva a rischio la conoscibilità da parte dell'imputato dei capi di imputazione contestati e la rettifica di questa impostazione è stata attuata. Dicevo all'inizio che il *corpus iuris* di cui ci stiamo occupando riguarda anche l'inasprimento dei reati contro il patrimonio ed è trattato dagli articoli dal 4 al 6 del disegno di legge.

Anche per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, regolato dall'articolo 3 del disegno di legge, è previsto un inasprimento del quadro sanzionatorio.

Veniamo ora a un altro delicato tema trattato dal disegno di legge: la delega per la riforma delle intercettazioni, che riguarda l'articolo 35. In questo articolo viene sviluppata la garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Si precisa la scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettato, nel rispetto del contraddittorio e delle esigenze di indagine. Viene dedicato uno speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a quattro anni, viene introdotta per punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, semplificato l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

ma con specifica motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato. Credo di aver superato il tempo a mia disposizione di trentatré secondi e, quindi, se il Presidente me le consente, continuo fino alla fine con altri due minuti e non di più;

delega il Governo a prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; a prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; inoltre la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e i limiti di proponibilità. Da ultimo, l'articolo 36 del disegno di legge prevede una semplificazione delle procedure: vi è la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, a eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. prevedono la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia la valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato; infine, l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario; un provvedimento per molti versi estremamente complesso, frutto di un serrato lavoro della Commissione giustizia, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo. Ricordando brevemente la gestazione di questo disegno di legge, come ha fatto nella relazione all'Assemblea il senatore Cucca prima della pausa estiva, la Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altri numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

esempio - autorevoli personalità come il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino; il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane. Il testo unificato, elaborato dai relatori e adottato dalla Commissione lo scorso maggio, ha assorbito anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge n. 1844, che tuttavia conteneva non pochi profili problematici.

per ricondurre alcuni aspetti critici ai criteri di ragionevolezza e rispetto delle garanzie e delle tutele insite nel principio dell'equo processo. Scopo principale di questo provvedimento è stato fin dall'inizio modernizzare il sistema giudiziario e rispondere alle esigenze rappresentate per un sistema moderno ed efficiente non solo dall'Unione europea, dagli operatori del settore e dalle commissioni ministeriali di studio che si sono adoperate per elaborare proposte di riforma e innovazione. Passando al merito del provvedimento, mi preme sottolineare come esso detti una disciplina innovativa riguardo alle intercettazioni: la delega al Governo prevede che sia garantita la riservatezza delle comunicazioni, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Si delinea un nuovo reato, per punire coloro che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate abusivamente per denigrare altre persone. non con positività si enuncia il principio della semplificazione dell'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Vengono precisamente delineati, infine, i limiti per l'utilizzo di captatori da remoto in dispositivi portatili, cioè registrazioni a distanza con *virus* *trojan*. I principi e i criteri direttivi per l'uso di questo particolare e delicato strumento sono stati formulati prevedendo che l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice, prevedendo come regola generale che il *virus* possa essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato prevedendo, infine, che i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale). Inoltre, ricordo come si intervenga positivamente per inasprire le pene di odiosi reati contro il patrimonio. L'articolo 4, infatti, interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale, che reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 euro a 1.032 Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 927 euro a 1.500 euro. L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali della pena sia detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) che pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali 2.065 euro a 2.500 euro, nel massimo). Vorrei quindi brevemente commentare gli altri punti cardine del provvedimento. Si è molto parlato negli ultimi anni di semplificazione delle procedure del processo penale: questo disegno di legge mira proprio a questo obiettivo quando detta norme di riforma dei giudizi di impugnazione. In particolare, mi riferisco a previsioni come la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; alla possibilità, per il procuratore generale presso la corte di appello, di appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; infine alla possibilità, per il pubblico ministero, di appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Vorrei ricordare la norma che prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di processi, che assorbono risorse economiche e strumentali, a essere celebrati con una semplicità e una soddisfazione di giustizia oggi impossibile. Questa opzione sarà prevista, ovviamente, per reati che non provocano allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa; e quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta. Il provvedimento dedica poi una specifica delega alla riforma dell'ordinamento penitenziario, al fine di implementare finalmente i principi della funzione rieducativa della pena e del rispetto della dignità delle persone detenute in carcere (uomini, donne e minori). Nello specifico, richiamo le disposizioni che incoraggiano all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui appunto si intende facilitare l'utilizzabilità; all'individuazione di attività di giustizia riparativa; alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. In questo quadro si è inteso attribuire dignità legislativa, secondo noi in modo virtuoso e attento alle istanze che tutti i giorni provengono dal nostro sistema penitenziario relativamente alle esigenze dei detenuti minorenni, nel senso di un maggiore accesso all'istruzione, alla crescita personale e sociale e ai bisogni particolari e specifici delle donne recluse e delle detenute madri, che vivono situazioni e realtà troppo spesso incompatibili con le loro condizioni. La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri. riforma della prescrizione, finalmente equilibrata, come votata dalla Commissione giustizia di questo Senato, dopo mesi di valutazioni e proposte differenti, alcune anche caratterizzate da profili di scarso garantismo liberale. Nello specifico, l'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo l'istituto rimane caratterizzato da un approccio liberale e garantista, ispirato ai principi dell'equo processo e di tutela del diritto alla difesa. In altre parole si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, il calcolo della prescrizione viene modificato per alcuni reati gravi di corruzione. Quindi, inserendo un ulteriore comma all'articolo del codice, si stabilisce che, per i reati di maltrattamenti in famiglia

salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Sul fronte del procedimento penale, vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse. Il testo contiene ulteriori importanti modifiche in questo settore, come gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. La Commissione, durante il proprio lavoro in sede referente, ha opportunamente concordato di rimandare a una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni; la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati. Il Gruppo di Area Popolare ha mantenuto in questi mesi un approccio costruttivo e di apertura al confronto con le altre forze politiche di maggioranza e di opposizione. Siamo convinti, infatti, che questo sia un provvedimento che porti innovazione, efficientamento e razionalizzazione all'interno di una macchina giudiziaria e penitenziaria che ha bisogno di maggiore attenzione da parte del legislatore. I nostri sforzi e le nostre proposte hanno sempre riguardato il merito del provvedimento, senza mai assumere contorni di arroccamenti preconcetti o inutilmente estremistici. In conclusione, mi sembra doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi della Commissione giustizia, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro contributo hanno consentito l'approvazione del testo che è stato portato in Aula. Un ringraziamento va rivolto anche al Governo, rappresentato dai sottosegretari Migliore e Chiavaroli

Signor Presidente, mentre dalle aule civili e penali della nostra Nazione sale l'implorazione da parte degli operatori di giustizia di cercare di frenare - o quantomeno coordinare - la produzione legislativa bulimica

su molti articoli del codice penale, del codice di procedura penale e addirittura sull'ordinamento penitenziario. Si tradisce, quindi, una chiara volontà chiara volontà di azione politica che sembra muoversi verso l'ormai annosa e censurabile prassi a cui facevo riferimento, ovvero una produzione legislativa disordinata, scollegata, disorganica, che non fa altro che rendere il quadro normativo spesso più confuso e certamente muovendosi lontano lontano da quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di una giustizia più efficiente e più giusta. Con questa breve premessa vado a esporre alcuni punti - alcuni dei quali sono già stati oggetto di

mesi dopo la sentenza di primo grado e diciotto mesi dopo la sentenza di secondo grado - come un pannicello caldo, che certamente, statisticamente, potrà influire su un certo numero di procedimenti che non esauriranno il loro corso con una

della prescrizione, come disposto dall'articolo 161 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche,

tanti operatori del diritto, giuristi, magistrati e non - sarebbe necessario. Riteniamo infatti che, in tema di prescrizione, bisognerebbe stabilire una volta per tutte che, all'esito di una verifica dibattimentale, dove l'esercizio di difesa si è potuto esplicare completamente, in caso di sentenza di condanna,

economici, psicologici, di equilibri familiari, di lavoro. Ecco perché mi piace ricordare che nelle nostre proposte emendative, dalla legge di stabilità fino al provvedimento che ci occupa, accompagniamo

Ciò vuol dire destinare anzitutto una somma superiore all'1,3 per cento del PIL, che oggi l'Italia riesce a destinare alla macchina giustizia; avere il coraggio di prendere decisioni storiche volte a migliorare le risorse umane, strumentali, logistiche e poi anche ordinamentali, per far sì che il diritto di avere una sentenza di assoluzione o di condanna - diritto dell'imputato e della collettività - sia garantito in termini ragionevoli e di equilibrio.

calerà su questo testo di legge così com'è o come modificato in un maxiemendamento. Con una cappa allucinante e insopportabile, su una materia così delicata come quella penale, il Governo

fatto riferimento è la delega che il Governo ritiene di doversi far attribuire in materia di intercettazioni.

Noi continuiamo a dire che non vediamo alcuna necessità di un intervento legislativo, tanto più fatto con delega e, quindi, con una formulazione che rischia di essere una norma in bianco, che metterà le mani

al diritto e all'efficacia dell'investigazione, al diritto alla difesa, che va sempre tenuto presente, e anche al diritto della *privacy* degli imputati e delle persone estranee. In quei protocolli, infatti, è previsto un sistema di tutela anche delle persone estranee ai procedimenti penali. Come

una norma che molti studiosi della comunicazione della rete, giornalisti, intellettuali e professori universitari già ci segnalano come estremamente pericolosa. Ben lungi dal voler tutelare le ragioni dei minorenni

qualora ritenuta diffamante e quindi lesiva della reputazione e dell'immagine altrui, se acquisita, dice il testo, fraudolentemente - è un avverbio dai contorni non molto nitidi,

in un video, in caso di diffusione, potrà tutelare il proprio presunto diritto sottoponendosi al rischio di un procedimento penale. E ciò avverrà con una sanzione penale davvero rilevante per questo reato, e noi sappiamo benissimo che ad oggi ancora c'è ed è vigente il reato di diffamazione, e non si vede la necessità di una tutela ulteriore, se non relativa, perché sono esclusi giornalisti, il diritto di cronaca o di difesa o nell'ambito giudiziario amministrativo. A chi si rivolge allora questa norma? Si rivolge al cittadino comune, e a noi piace pensare ai nostri concittadini, attivisti o no, del Movimento 5 Stelle, a coloro che sono ancora costretti a entrare nei consigli comunali - per esempio - dove vigono regolamenti che non permettono le riprese video di quella che dovrebbe essere la casa trasparente dei cittadini del Comune. del Comune. Questa norma potrà allora essere utilizzata da un consigliere comunale che, ritenendosi leso nella propria reputazione e immagine perché ripreso da un cittadino presente nel pubblico, che poi magari ha diffuso anche parte di un di un suo intervento in Aula, potrà denunciarlo lamentando questo tipo di lesione. Questa norma liberticida, inutile perché la tutela della *privacy* e della propria reputazione già esiste, accompagnata con quanto ci sta per arrivare dalla Camera,

della rete o delle persone, della testa di tanti nostri connazionali, che non deve avere nulla a che fare con la neutralità e la libertà di pensiero e di libertà di pensiero e di espressione che si deve poter svolgere in quello che è l'unico mezzo che ancora, bene o male, garantisce una libertà dai grandi gruppi editoriali o dalle linee politiche imposte da qualcuno. Vedo che

magari in un'ottica di difesa contro il «giustizialismo» che può affiorare, abbia speso una parola su quanto previsto nell'articolo 33 in in tema di partecipazione a distanza all'udienza. Si tratta delle videoconferenze che, nel testo di legge disposto, sono stabilite di ufficio, automaticamente dal giudice senza alcuna possibilità di valutare casi per una serie di reati. reati. Capiamo benissimo: è una norma comprensibile, volta al risparmio dovuto alla mancata traduzione di persone detenute in un'altra città. In tal caso va bene che l'esame di un imputato o anche di un testimone possa svolgersi in videoconferenza, consapevoli, per chi

difesa. Si dice che in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo a distanza, il giudice, su istanza, può consentire alle altri parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. Si dice che se gli avvocati e le parti ulteriori rispetto all'imputato o agli imputati - quindi possiamo pensare alle parti civili o agli imputati per reato connesso e a tutta una serie di figure processuali - vogliono partecipare alla videoconferenza, devono farsi

La settimana scorsa abbiamo tutti letto la triste notizia del primo ufficiale donna arrestato a Taranto in esito a fatti di corruzione, fatti dei quali si è venuti a conoscenza mediante l'utilizzo dei *trojan*, che consentono di azionare a distanza il microfono di un cellulare per potere acquisire prove e fonti informative che possono verificare o no la consumazione di un reato, magari contro la pubblica amministrazione. Segnaliamo - e abbiamo all'uopo presentato emendamenti abrogativi o sostitutivi - che aver disposto nel testo attuale che questa modalità possa essere attivata

indubitabilmente, non farà altro che limitare la capacità investigativa. Essa presupporrà, infatti, un controllo preventivo, o anche di utilizzabilità *a posteriori*,

Sarebbe evidentemente più ragionevole prevedere che alle Forze dell'ordine, nei casi previsti e con i limiti imposti - nessuno pensa alla pesca a strascico e a una intercettazione collettiva, tantomeno noi e speriamo neanche voi

Signor Presidente, quando si parla di giustizia, il tema è talmente complesso, articolato

ha portato a un risultato veramente molto equilibrato e anche molto saggio. So perfettamente che la mia posizione sulla giustizia non è uguale a quella del collega Casson. Eppure, con il collega Casson ci siamo confrontati e abbiamo trovato un punto di raccordo, sempre per un fine migliorativo. So che continueremo ad avere posizioni diverse e che il senatore Casson continuerà a sostenerle, così come continueremo a sostenere la bontà di questo testo il mio Gruppo

suoi componenti, il Governo, nella figura del sottosegretario Chiavaroli, i Capigruppo di maggioranza e di opposizione, lo stesso relatore e il presidente D'Ascola se il testo che noi andremo ad approvare ha una sua *ratio* e un suo equilibrio, che noi vorremmo mantenere

anche a un lavoro serrato di confronto su temi - ripeto - estremamente complessi e articolati. Devo dire che la saggezza del sapersi fermare a un certo punto e, per un bene maggiore, rinunciare anche a una posizione precisa, puntuale, nella quale si crede è un valore che io ritengo estremamente positivo e del quale voglio rendere anche merito al collega Lumia,

caso il bene superiore non contrasta certamente con le posizioni che possono essere di tipo personale o di cultura o di appartenenza.

è frutto di un confronto serrato tra posizioni diverse (la ricchezza della politica sta anche in questo confronto serrato e spesso aspro, ma che ha come fine ultimo, soprattutto in un campo così delicato come quello della giustizia, il bene dei nostri cittadini). Signor Presidente, io leggerò alcune parti del mio intervento, poi le chiederò la cortesia di poterlo pubblicare

Il provvedimento in discussione oggi in Aula si pone come una riforma globale e complessiva del processo penale. Le finalità sono molteplici: *in primis*, uno degli obiettivi principali è la diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, che si pone in modo contestuale al potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale. Il potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese viene raggiunto anche attraverso il rafforzamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale. Inoltre, l'ammodernamento della disciplina dell'infermità mentale, e il potenziamento degli effetti rieducativi dell'esecuzione penale sono due degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del sistema penale come emerso dalla laboriosa attività della Commissione giustizia. Obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti con tenacia e faticosi compromessi. Vorrei dire che quando si parla di compromessi si pensa sempre che siano al ribasso, mi chiedo però perché non possiamo invece pensare di aver fatto dei compromessi al rialzo, cioè di aver portato delle novità e delle positività nel processo penale. L'obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è raggiunto, nell'ottica della riduzione dell'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato: tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l'adozione da parte del reo di condotte riparatorie, in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale. Ulteriore strumento è la delega al Governo per l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata ed ai reati contro il patrimonio. Nell'ottica di limitare la durata dei procedimenti penali, evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pena anticipata per l'imputato, si muovono poi le modifiche al codice di procedura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari, a garanzia dell'indagato, sia del processo, in particolare, ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento; limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza, in caso di giudizio abbreviato; soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari e, soprattutto, della Corte di cassazione. In particolare, la riforma dei giudizi di impugnazione prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d'appello di appellare soltanto nei casi di avocazione e acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». L'obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento della centralità del reo nel processo penale e di correlativa maggiore attenzione alla vittima, vuole essere rafforzato attraverso modifiche al codice di procedura penale che garantiscono il diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari, nonché la previsione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla alla persona offesa della richiesta di archiviazione, ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa. Nel senso del potenziamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale si muovono, poi, le deleghe al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (soprattutto al fine di adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione di protezione dei dati personali) e per una nuova disciplina delle intercettazioni. Quest'ultima si dovrà ispirare a principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare, quelle non rilevanti o relative alle persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento: sappiamo molto bene come

punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l'immagine altrui. In tale settore il lavoro della Commissione ha portato alla disciplina dell'uso dei captatori informatici, cosiddetti *virus* Trojan: al fine di consentirne un impiego efficace e allo stesso tempo rispettoso della *privacy* dei cittadini, l'utilizzo di questo strumento rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato. In particolare, i Trojan potranno essere impiegati nel quadro di una disciplina governativa che dovrà prevedere che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; quindi, al termine della registrazione il captatore informatico dovrà essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile; dovranno essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale, per garantire che il *virus* si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. Inoltre, fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero potrà disporre tale tipo di intercettazioni, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. Infine, si dovrà prevedere che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede. Sul tema della prescrizione, il compromesso raggiunto durante i serrati lavori della 2a Commissione consiste nella sospensione della decorrenza della prescrizione pari ad un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo, a nostro parere, vengono soddisfatte esigenze di duplice profilo: da una parte l'esigenza processuale di tempi più lunghi per celebrare tutte le fasi procedimentali, dall'altra quella di mantenere la natura garantista dell'istituto, a tutela dell'imputato. È stata sicuramente migliorata la disciplina contenuta nel precedente disegno di legge n. 1844, proveniente dalla Camera e quindi confluita nel testo unificato che ha esaminato e approvato la Commissione giustizia del Senato. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto un regime di stampo liberale, equilibrato, seppure con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini, per le fasi di impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso Signor Presidente, vorrei soffermarmi, in particolare, su un aspetto che a mio avviso risulta particolarmente innovativo e che nel trambusto mediatico sulla prescrizione è passato leggermente in secondo piano. Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri. La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri. Di particolare rilievo la previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica. La disciplina di specifici interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri permette in tal senso la possibilità per le donne di vivere la loro maternità, nonostante la momentanea privazione della libertà. Di particolare rilievo ed interesse sono i principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età. Nello specifico si prevede una giurisdizione specializzata

la previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; la previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni. Tutti questi principi orienteranno l'azione riformatrice del Governo nell'attuazione di un ordinamento penitenziario efficiente e moderno. Continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo si parla della lunghezza del processo in tutti i *talk show* e in tutte le conferenze, quando puntualmente si segnalano i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese a livello economico e di credibilità internazionale. Quindi, rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre di mali cronici che tutti ben conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Questo provvedimento apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, colleghi della Commissione giustizia con i quali abbiamo lavorato a lungo su questo provvedimento, collega Chiavaroli che ha rappresentato bene il Governo durante questo lavoro, ci troviamo oggi a esaminare, semplicemente leggendo il titolo della nota breve in distribuzione, «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario». Credo che sia il caso di soffermarci, all'inizio di un breve ragionamento che vorrò fare, su cosa sia il processo penale. Sapete che il nostro codice ha subito una recente

una complessiva riforma del processo penale introducendo il sistema accusatorio. Per definire, dal punto di visto storico, ma anche direi giuridico e politico, che cos'è il processo penale nel nostro Paese,

il processo non tanto è un giudizio quanto si compone di una moltitudine di giudizi,» - poi torneremo su questo richiamo alla moltitudine dei giudizi - «delle parti, dei testimoni, dei consulenti e del giudice, l'ultimo dei quali, in ragione dell'autorità di chi lo ha emesso, ha un'efficacia particolare, ma a considerarlo attentamente scopriamo come esso sia una regola di condotta, ossia una norma, poiché il giudice quando sentenzia comanda. Senonché il comando esce da una trama di operazioni logiche regolate dal diritto ed ecco un groviglio di atteggiamenti, rituali, logici, normativi». Penso che queste poche righe, che qualsiasi studente di diritto in questo Paese può attingere da questo meraviglioso manuale, siano una giusta guida anche per anche per noi che abbiamo fatto un grande lavoro nel tentare una riforma corretta, conferendo poi ovviamente anche una delega al Governo, sul processo penale. Per questo torniamo

dai fatti recenti e da come spesso sono stati narrati dai giornali, emerge che il processo questo non è, ma in realtà noi dobbiamo essere ligi alle nostre regole e sapere che esiste,

e condanne già scritte dai titoli dei giornali quando alcuni procedimenti penali sono solo all'inizio, ai primi passi, ma su questo tornerò. considerazione serve a capire che abbiamo fatto un grande lavoro di riforma e di approfondimento e questo Governo certamente, attraverso l'opera esimia e fantastica del ministro Orlando, è l'Esecutivo che sta facendo di più in in termini di riforma del processo, in particolare del processo penale e di tutto quello che ne promana. Pensate a che senso e che significato, prima di tutto umano, ha avuto il lavoro che abbiamo svolto sull'esecuzione della sentenza penale con i tre giorni degli Stati generali dell'esecuzione penale, lavorando all'interno di un carcere e lavorando proprio su quello che è poi l'esito finale

con un ordinamento penitenziario che non garantisce fino in fondo che la pena sia rieducativa e su questo ancora abbiamo molto da lavorare. A questo punto, con questo testo abbiamo cercato di dare efficienza ad un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. Infatti è chiaro a tutti noi, e lo vediamo quotidianamente, che il malfunzionamento del sistema giudiziario è uno dei macigni più grandi

europei. Entro brevemente nel merito: quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali, ma che è anche di diritto sostanziale. Certamente vale brevemente la pena di ricordare l'impianto del testo su cui abbiamo lavorato in Commissione. Prima di tutto abbiamo lavorato sull'estinzione del reato, sulle condotte riparatorie e su modifiche ai limiti della pena per i delitti di scambio elettorale politico‑mafioso, furto e rapina. una delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Abbiamo poi modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, nonché modifiche molto importanti in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale, struttura della sentenza di merito e semplificazione delle impugnazioni. Per quanto riguarda la semplificazione delle impugnazioni, noi giochiamo una carta importantissima: ci giochiamo, la vera capacità di incidere verso quel grande principio fissato da tutte le norme in materia di giusto processo: un giusto processo è giusto quando è breve, è giusto quando il cittadino sottoposto se condannato, vede la sua condanna emanata in tempi brevi e certi, e può espiare la pena alla quale è stato condannato con rispetto dei suoi diritti umani. Quindi l'aver interloquito - e secondo me su questo c'è anche materia per andare avanti sul secondo e sul terzo grado, cioè sull'appello e ricorso per Cassazione - dà già un segno di dove noi vogliamo arrivare. Probabilmente sarà giusto arrivare, non dico all'estinzione completa, ma ad un parziale asciugamento - molto stretto - dei motivi di ricorso in Cassazione e limitare ancor di più al vizio di legittimità tranne casi tranne casi particolari, il ricorso per Cassazione. Noi su questo abbiamo certamente materia per andare avanti e per andare avanti bene. Infine, la delega al Governo tocca la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Ho sentito alcuni interventi di altri colleghi e proprio per questo voglio specificare che noi siamo intervenuti con efficacia su alcune previsioni. Pensate all'aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico‑mafioso, proposto nell'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione, che prevede la reclusione da sei a dodici anni, in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per il reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, specie per la previsione di cui al primo comma, alla quale è stato per molti anni espressamente agganciato. Va peraltro tenuto presente che nel 2015 la pena per il reato di associazione mafiosa è aumentata, prevedendo,

lezione in termini di repressione dei reati collegati alla mafia e ad altre criminalità. Siamo intervenuti inoltre sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva da uno a tre anni ed abbiamo inasprito il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma Siamo anche intervenuti sull'articolo 625 (l'articolo seguente del codice penale), che elenca le circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, inasprendo il quadro sanzionatorio e prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni. Anche questa è una risposta concreta e reale al diffuso senso di insicurezza, che qualcuno ritiene di impunità, nei confronti di certi reati che ampliano l'allarme sociale. Ma è solo questa la risposta concreta: guai a fomentare, guai a sostenere, guai a in qualche modo posizioni pericolose di chi si vuole fare giustizia da solo o di chi inventa altri meccanismi al di là del giudizio e del codice penale. Quindi è giusto l'inasprimento delle pene, in un ambito più più ampio di repressione dei reati che creano incertezza sociale. Andando avanti, torniamo al punto che io ritenevo molto importante, quello della semplificazione Le impugnazioni saranno quindi semplificate, i motivi di appello andranno ad un vaglio più rigoroso e vi sarà un effetto deflattivo sui ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale abbiamo reintrodotto l'istituto del concordato sui motivi di appello. Su questo è stato detto poco. Credo invece che sia importante ribadire che il concordato sui motivi di appello consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, contestuale rinuncia ad altri eventuali motivi, facendo dunque salva, in ogni caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato, la possibilità di ordinare la citazione a comparire nel dibattimento. Vedete quindi che mai e poi mai la nostra intenzione è stata quella di legare le mani al magistrato. Nel corso dell'esame che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbiamo comunque introdotto alcune limitazioni significative. una su tutte: grazie all'approvazione di emendamenti del Partito Democratico, abbiamo approvato l'esclusione dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti per i procedimenti per cui ai delitti dell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3 e 3-*quater* del codice di procedura penale, per i delitti sessuali, per i delitti sessuali compiuti in danno a minori di età e infine per i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Parliamo di delitti odiosi, terribili, terribili, che hanno una pericolosità sociale molto alta, perciò abbiamo ritenuto di dover sottrarre da tale ambito...

ha fornito i numeri di questo orrore, informandoci che in Italia, ogni 2,2 giorni, viene uccisa una donna e che il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Poco si parla della violenza assistita, ma qual è la gravità che incombe sulla vita di un bambino che assiste continuamente a violenze nei confronti della propria madre, a maltrattamenti, a insulti, a insinuazioni, fino ad arrivare all'estremo evento della morte? Anche per questo motivo - e sarò breve, signor Presidente - abbiamo escluso ogni possibile accordo sui motivi di ricorso per questi orrendi reati.

quasi esclusivamente o solo ed esclusivamente nella testa degli uomini. Abbiamo un problema culturale nell'affrontare questo tipo di reato e ciò dovrà essere ribadito nei procedimenti e nelle pene. Purtroppo assistiamo ancora a troppe distrazioni, a maltrattatori che escono dal carcere con grande facilità

tutti quegli atti culturali tendenti alla valorizzazione delle discriminazioni piuttosto che alla loro condanna. È necessario, quindi, intervenire con la cultura nella scuole, affinché l'educazione alla differenza di genere, che include come ricchezza come valore ogni diversità, venga affermata presto. Bene ha fatto questo Governo, attraverso la nostra Ministra dell'istruzione, a dire che già da ottobre cominceremo a occuparci di differenza di genere nelle scuole. Concludo velocemente, signor Presidente,

Nessuno di noi vuole fermare strumenti di indagine, ma è impensabile che si proceda ancora allo sfruttamento di quelle che l'articolo 191 del nostro codice di procedura penale definisce prove inutilizzabili per dare per dare evidenza mediatica e alla vita privata di persone che, se responsabili, saranno condannate, ma non devono esserlo per l'uso, l'abuso e la strumentalizzazione

e, stamattina, il collega Mineo ha dato una ragione del nostro modo di comportarci, ha detto chiaramente che vi è uno scontro, all'interno della maggioranza, tra due filosofie che non emergono nel dibattito.

si tocca un sistema sanzionatorio che deve rispondere ad una razionalità; non può esserci uno squilibrio tra reati e reati, nella determinazione della pena, prescindendo dalla gravità, dalle persone coinvolte e

Le regole processuali servono ad assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione, una funzione che può svolgersi solo se le regole del processo sono calibrate sui principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e del nostro ordinamento giuridico. Certamente, come ha detto il senatore Mineo, vi è uno scontro all'interno della maggioranza tra chi prescinde da questi principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento e chi invece è costretto, per ragioni di equilibrio della maggioranza, ad adattarsi a partorire norme che sono liberticide, come dirò tra poco. Quando si stabiliscono le regole del processo, se si vuole garantire la vera funzione del processo, allora incominciamo col dire che l'iscrizione nel registro degli indagati deve avvenire nel momento in cui il pubblico ministero ha la notizia di reato e, se si vogliono realizzare l'effettiva tutela e l'effettiva garanzia dei diritti, deve iscrivere il nome reale di chi è indagato.

Abbiamo presentato questi emendamenti e se ne è discusso. Nonostante la Commissione abbia accolto 28 emendamenti del nostro Gruppo, su alcune questioni di fondo ha glissato.

con un'alta espressione, si definiva convergenza di interessi contrapposti per realizzare un prodotto legislativo che possa tener conto di tutti i diritti e gli interessi che possono esserci.

con molta correttezza. Il Ministro della giustizia ci ha fornito i dati in questa Assemblea, quando abbiamo discusso dei reati contro la pubblica amministrazione l'anno scorso e quando ne abbiamo discusso in Commissione. L'attuale tempo di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione non supera il 2 per cento. Anzi, in molti uffici giudiziari italiani è pari allo

processo. Prima di queste follie, la bancarotta era il tempo più lungo di prescrizione. Andate a vedere quanto duravano i processi per bancarotta rispetto agli altri. Noi abbiamo dato parere favorevole all'introduzione di un corsia privilegiata per i reati contro la pubblica amministrazione perché occorre individuare immediatamente se è responsabile un corrotto.

processo. Ho sentito il presidente Lumia che ha parlato di doppio binario e ha citato Falcone. Mi dispiace, Lumia, non citarlo. Non lo avrebbe mai fatto. Dopo la fine dell'indagine preliminare, quando il giudice, il pubblico Ministero, deve assumere solo la decisione

La collega Cirinnà ha fatto riferimento all'accordo tra le parti nel giudizio di appello;

un'indicazione secondo la quale il procuratore della Repubblica dovrebbe dare degli indirizzi ai vari sostituti per procedere al cosiddetto patteggiamento di appello. Tra gli elementi da valutare avete indicato la complessità del procedimento, come se in ragione della complessità e, quindi, dell'incapacità, a quel punto, del pubblico Ministero di sostenere la complessità, egli si accorda per una pena più bassa di quella che dovrebbe essere erogata. Vi rendete conto che ciò è assurdo?

Qual è la funzione della pena? È su quella che deve intervenire la valutazione ai fini dell'accordo. Io ho applicato questa norma quando vigeva nel nostro ordinamento, da magistrato e come sostituto procuratore generale della corte d'appello di Milano.

sentito dire poi che questo provvedimento porterà alla crescita economica. Scusatemi, se parliamo del processo civile, è un'altra questione;

sono condizionati dalla credibilità dell'istituzione, dalla credibilità dello Stato. Noi abbiamo sottoscritto vari accordi in sede comunitaria. Sento qui molti di voi appellarsi sempre all'Europa, alle grandi sensibilità del diritto comunitario, delle sentenze di Strasburgo, ma quando si tratta di applicarle, ve ne dimenticate. Alcuni di voi può darsi che non si ricordino che sette o otto anni fa fu approvata una norma in quest'Aula. È quella norma, che nei testi di diritto comunitario viene indicata come "legge Azzolini", recante l'obbligo per il Parlamento di valutare una relazione sullo stato di attuazione delle sentenze di Strasburgo nel nostro Paese. Sapete quante volte questa relazione è stata discussa dal Parlamento? Mai.

che io sono stato condannato in base a un reato inesistente, per cui nel nostro Paese si realizzano processi

Una di queste riguarda la sentenza contumaciale, nei confronti appunto del contumace, per cui, ora, l'appello deve ripetersi. E anche in questo provvedimento viene previsto specificamente che deve essere rinnovato l'esame istruttorio,

non cogliamo l'occasione per porre rimedio al problema della inesecuzione delle sentenze di Strasburgo. Come sapete, appena

o non faceva parte dei disegni di legge proposti qui dentro. Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Qual è la vostra idea di garanzia del diritto? Qual è la vostra idea di garanzia del più debole? Qual è la vostra idea di rispetto del diritto comunitario? Io sento tutti i giorni il senatore Lumia e altri colleghi parlare di Europa e di diritto comunitario. E poi? Vergogna! Quando si tratta di applicare una delle regole fondamentali del diritto comunitario, cioè il rispetto delle sentenze di Strasburgo, mi si dice che la mia proposta è inammissibile in questo provvedimento. Ma vi rendete conto? Qui stiamo parlando di processo penale!

un'arma nei confronti dell'avversario, nei confronti di colui che ha sbagliato. Io ho fatto per anni il pubblico ministero e non ho mai provato odio nei confronti di imputati contro i quali chiedevo anche l'ergastolo. È necessario necessario sempre il rispetto, anche di chi è condannato, perché al centro della nostra azione, al centro del nostro sistema giuridico, c'è la persona, con la sua dignità.

8, lettera *b)*, secondo periodo, quando si dice: «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere». Sono le

Se, per ipotesi, io mi trovo al processo di appello e sono trascorsi otto anni e dieci mesi, devo contare la sospensione? Se devo farlo e quindi pronunciarmi

Non dimenticate che quando sul falso in bilancio vi ho pregato di fare una precisazione sulle valutazioni perché altrimenti il dubbio interpretativo avrebbe determinato conseguenze negative,

sentendo quest'ultimo intervento mi è tornata in mente la legge sull'eterogenesi dei fini:

Il dibattito ha offerto anche altre pagine del cosiddetto "benaltrismo": è altro che va fatto; è altro che deve essere risolto. Senza mai indicare cosa sarebbe questo ben altro. ha anche portato delle dosi di "disfattismo" essenzialmente concentrate sul tema della prescrizione e delle intercettazioni,

e lo scambio elettorale politico-mafioso, all'estinzione del reato per condotte riparatorie (che è, credo, una misura di grande civiltà giuridica); dalle modifiche relative alle condizioni di improcedibilità per i reati con pene edittali detentive non superiori nel massimo a quattro anni (fatta eccezione per i reati contro il patrimonio e per il reato previsto dall'articolo alle modifiche relative al casellario giudiziario; per non parlare delle modifiche riguardanti le indagini preliminari, il provvedimento di archiviazione, l'appello e il ricorso in Cassazione e la rescissione del giudicato, istituto a garanzia del diritto di difesa. Credo sia molto importante e che meritasse un approfondimento e un'attenzione la riforma dell'ordinamento giudiziario. Penso a tutte le norme sulle misure alternative: la revisione dei presupposti di accesso, l'osservazione scientifica della personalità del reo, la maggiore efficacia dei controlli, l'eliminazione degli automatismi ostativi all'individuazione del trattamento rieducativo e alle differenziazioni dei percorsi penitenziari, le misure di giustizia riparativa quali elementi fondanti del percorso di recupero sociale, l'incremento della forma di lavoro retribuito, delle forme di volontariato del detenuto e del reinserimento dei condannati, la valorizzazione del diritto all'affettività, l'integrazione dei detenuti stranieri, la responsabilizzazione dei detenuti e la libertà di scelta. Questi sono tutti criteri sono tutti criteri di delega che dimostrano quanta attenzione si pone, in modo decisivo, e - spero - anche innovativo (ce lo dirà il decreto legislativo), sulla rieducazione della pena e

sono il miglioramento della personalità e la proiezione oltre il carcere, e si rischia di portare il carcerato, al momento della fine della sua detenzione, a diventare una persona che non ha più motivazioni, capacità e forza per reinserirsi nella società. Credo che non meno importanti siano le misure misure di riforma dell'ordinamento penitenziario riguardanti i minori. Mi riferisco alla sottolineatura dell'esigenza di fare molta attenzione alla socializzazione, alla responsabilizzazione, alla promozione e alla crescita della persona.

di un trattamento e una cura che, per il giovane adulto, non possono non avere una soluzione di continuità con quelle avuta fino al giorno prima. L'ampliamento delle misure alternative con l'ampliamento delle forme di affidamento ai servizi sociali e della semilibertà: tutto questo rientra fortemente nell'ottica della rieducazione, dell'aggancio con la società del domani, del dopo pena.

alle madri sottoposte a misure cautelari del diritto alla misura alternativa per poter allattare e curare i bambini di minore età. Questi non sono interventi marginali. Penso che tutto ciò, nella logica dell'articolo 27 della Costituzione, introduca princìpi idonei a rafforzare, quando non ad introdurre, strumenti e condizioni di vera

intercettazioni. Si grida al bavaglio, alla violazione del diritto di cronaca e della libertà di espressione: chi vuole lo Stato poliziesco o un modello di Stato contrario ai fondamenti dello Stato liberale e democratico può sostenere questo; chi è garantista e non giustizialista non può che rigettare simili accuse. Con queste misure infatti si perimetra l'uso delle intercettazioni giudiziarie che, proprio perché tali, non possono che essere usate solo ai fini di giustizia. Si impedisce - per essere ancora più chiari - di avallare la prassi, indegna di uno Stato di diritto, del processo mediatico e del processo extragiudiziario per fatti non costituenti reati, ma accertati nel corso di indagini penali. Si impedisce che si consolidi un circuito mediatico‑giudiziario, credo involontario per molta parte, che al di fuori delle garanzie del contesto alimenti la caccia alle streghe. I diritti delle persone, quelli degli articoli 2 e 3 della Costituzione, vengono sempre prima e la loro tutela non comporta sconti alle responsabilità e alla punizione degli illeciti, ma impedisce, deve impedire, gli abusi di ogni tipo e di ogni genere. cosa stabilisce la delega sulle intercettazioni? In relazione all'articolo 15 della Costituzione, cioè il tema della segretezza della corrispondenza, fissa la garanzia della riservatezza dei colloqui difensori‑assistiti. Se qualcuno ha dei dubbi sulla costituzionalità di questa misura, legga gentilmente l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, ossia il diritto inviolabile della difesa.

Vorrei solo ricordare gli articoli 2 e 3 della Costituzione, i diritti inviolabili della persona, che sono più che mai pieni non si trova nella situazione di avere indagini di natura penale. o contenenti dati sensibili o dati che non siano pertinenti per i reati per cui si procede o per altri. Questa norma è contro giustizia? Io credo che sia in linea con il senso di giustizia nel modo più pieno. Quanto al divieto di trascrizione sommaria delle intercettazioni, perché contestare una misura di questa natura? La trascrizione sommaria non è la rappresentazione notarile di ciò che l'intercettazione ha consentito di appurare, ma è un'interpretazione dell'intercettazione. È forse contrario alle esigenze di giustizia vietare la trascrizione sommaria, cioè un'interpretazione del dato della trascrizione? Le prove, come principio generale, sono soggette al solo apprezzamento del giudice. E dunque? È previsto il delitto per la pubblicazione di audiovisivi e di registrazioni fraudolente che sia voluta al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui. È forse questo un limite alla libertà di espressione o è forse questo una tutela dei diritti delle persone? Vorrei che i tragici fatti a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni ci ricordassero quanto è sacrosanta anche una norma di questa natura.

sia una delega puntuale e che abbia principi che sono già precetti e che quindi, sotto questo profilo, abbia davvero, in modo più tangibile di altre deleghe che abbiamo votato, i caratteri propri della delega così come costituzionalmente definita. Con queste norme non c'è alcun bavaglio, alcun limite alla funzione giurisdizionale, la quale deve tradursi, finalizzarsi e limitarsi alla *iurisdictio*. Ma c'è casomai la più chiara responsabilizzazione nell'uso delle intercettazioni. Veniamo alla prescrizione: la prescrizione è una previsione necessaria per la certezza del diritto, della punizione e dei diritti della persona sottoposta a processo, diritti che non sono annullati da un rinvio a giudizio o da un avviso di garanzia. Chi ha sbagliato deve essere chiamato a rispondere, ma non può essere tenuto *sub iudice* per tempi indefiniti. Basta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo per dare la risposta alle visioni giustizialiste o dello Stato di polizia o di un'eterna condizione di indagato. La prescrizione, peraltro, è una misura, in termini di teoria generale, a tutela del soggetto passivo di un rapporto per evitare l'abuso del diritto rappresentato dal non esercizio dello stesso in funzione di tenere in scacco il soggetto passivo. La prescrizione non può essere a copertura delle inefficienze della macchina giudiziaria. Così si può giustificare una misura, come quella odierna, solo perché legata, se legata, a un progetto di riorganizzazione e di riforma dei tempi della giustizia. Un problema che chiama a una piena responsabilizzazione la magistratura, oltre agli altri soggetti del sistema, perché i ritardi in taluni casi indegni di un Paese civile non sono un problema e una colpa solo degli altri attori della giustizia, dello Stato o del legislatore. I ritardi chiamano in prima linea anche i magistrati stessi. Lo dimostrano i casi in cui Presidenti illuminati hanno eliminato gli arretrati e ridotto i termini dei processi senza norme straordinarie e lavorando sulla riorganizzazione degli uffici e sui tempi di lavoro. In un quadro ovviamente più complessivo e organico continuo a pensare che la responsabilizzazione legale dei giudici sui tempi del giudizio non leda né autonomia né indipendenza, ma costituisca un'applicazione della ragionevole durata del processo. Mi auguro che giungano segni concreti su questo piano, convinto che misure diverse, quali i limiti del diritto di azione, per quanto oggi necessarie come misure

per quanto riguarda le modifiche della prescrizione, vorrei osservare che c'è forse qualcuno che pensa che prevedere per i reati sessuali e pornografici - articolo 392, nei confronti di minori che la decorrenza della prescrizione parta dal giorno del compimento dei diciotto anni della vittima sia una misura ingiusta? Davvero si crede che l'aumento dei limiti della prescrizione, portata da un quarto a un mezzo, sia così decisiva? Rimangono i diciotto mesi di sospensione tra primo e secondo grado e i diciotto mesi tra il secondo grado e la sentenza definitiva. Sono una misura forte, non auspicabile ma comprensibile per lo stato della giustizia. Appunto. Per lo stato della giustizia che, nonostante gli sforzi del Governo e del ministro Orlando, rimane un problema e una sfida che questo Governo ha ancora il tempo e la forza di poter affrontare. Da cittadino mi auguro che ciò avvenga.

anche in considerazione dei toni pacati che quasi tutti hanno utilizzato. Sono stati offerti spunti di riflessione abbastanza complessi. Gli argomenti sono delicati e, per qualche

Roma ha circa 2.864.000 abitanti. Gli aventi diritto al voto sono 2.363.776. All'ultima elezione hanno votato 1.347.352 cittadini.

Ovviamente, democraticamente, la sindaca eletta, insieme ai suoi consiglieri, ha l'onere e l'onore, anche attraverso la sua Giunta incompiuta di Governo, di governare Roma,

oggi, noi del Gruppo Italia dei valori, ci domandiamo e domandiamo alla sindaca se sia stata fatta un'effettiva valutazione urbanistica del caso da parte dell'assessore, una valutazione che rilevi se Roma città eterna, imperiale, olimpica, sia in grado di supportare e sopportare un simile evento. La motivazione addotta a giustificare il «no» - e noi di Italia dei Valori pensiamo l'opposto, ovviamente - si riduce a due questioni. le Olimpiadi creerebbero maggior indebitamento: sarebbe opportuna in proposito una precisa valutazione da parte dell'assessore al bilancio, non pervenuta. In secondo luogo, potrebbero moltiplicarsi i fenomeni di male pratiche e corruzione durante i lavori di adeguamento delle strutture ricettive coinvolte nei giochi olimpici. Ora, una forza che governa ha l'onere di mettere in atto tutte quelle buone pratiche e quei controlli che prevengano il malaffare e non ha il diritto di sottrarsi dal mettere in atto investimenti che, se ben gestiti, possono mettere in moto un circolo virtuoso a vantaggio della città e della nazione. Il punto è saper gestire e saper governare i processi messi in atto. Ciò è possibile se chi governa ha capacità di sapere: saper fare, saper essere, saper divenire. Non è sufficiente proclamarsi onesti. Onestà fa rima con capacità, ma non significa esserlo. La capacità governativa la si dimostra attraverso azioni e sfide, anche difficili, come le Olimpiadi. Se si hanno le capacità, si riesce a prendere in carico grandi oneri, dimostrando di riuscire a fare, rimanendo onesti ed operando nella legalità. Avere rinunciato alle Olimpiadi per soddisfare un grillo nella testa fa pensare ad una mancanza di democrazia partecipata, tanto sbandierata e poco perorata: una mancanza di decisioni condivise democraticamente. Ma soprattutto fa pensare che chi è alla guida della Città eterna non ha piena contezza di cosa significhi governare Roma. Noi di Italia dei Valori sosteniamo le ragioni di Malagò

grazie